da notizie di stampa di oggi so aver già iniziato delle attività di accertamento, perché svolga al più presto una sommaria verifica di questa vicenda e riferisca in Aula, trattandosi di una questione che non ha risvolti solo locali, ma nazionali e che, forse, vanno anche al di là del territorio nazionale. La popolazione è molto, molto preoccupata e vorrebbe conoscere i provvedimenti immediati per limitare al minimo o eliminare - speriamo - nel tempo i danni derivanti da questa situazione di gravissimo pericolo ambientale. intervento. Naturalmente, non mi era sfuggita la presenza nella nostra Regione di questo enorme problema,

Si è giunti alla fase della replica, ma, inspiegabilmente, non sono stati espressi i pareri rispetto agli ordini del giorno presentati. Le chiedo, Presidente, se non sia il caso, visto che la risoluzione era finalizzata al Vertice di Berlino del

Signor Presidente, onorevoli senatori, gli obblighi al rispetto di vincoli comunitari sono alla base della necessità e urgenza del provvedimento di cui l'Aula del Senato di occupa. Un provvedimento che propone contenuti fra loro indubbiamente eterogenei, ma accomunati dal comune proposito di dare urgenti risposte a impegni di fonte sovranazionale, per porre termine a diversi contenziosi già in atto in sede comunitaria. È il caso previsto dall'articolo 1, per il quale va evidenziato che il contenzioso comunitario legato agli aiuti concessi dallo Stato alle società cosiddette ex municipalizzate è giunto a un al livello di assoluta urgenza. Il comma 1 dell'articolo 1, appunto, dà attuazione alla decisione della Commissione europea, che aveva riconosciuta come aiuti di Stato l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (l'IRPEG ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria La finalità di questo articolo 1 è appunto quella di porre fine al contenzioso pendente tra la Repubblica italiana e la Commissione europea. In particolare, al comma 1, si dispone per che sia attribuita all'Agenzia delle entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatesi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito. Il comma 2 autorizza l'Agenzia dell'entrate a liquidare gli importi, le imposte con i relativi interessi, da restituire all'amministrazione finanziaria.

In questo modo si definiscono e procedure con cui si procederà agli adempimenti. Restano escluse dall'iscrizione al ruolo automatica le posizioni il cui importo oggetto di recupero rientra nei limiti delle regole definite, cosiddette del *de minimis*, come indicato nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1. Le società che intendono avvalersi di tale regolamentazione, si dispone al comma 9, dovranno produrre apposita

di specifiche audizioni attraverso le quali si è potuto acquisire il quadro della platea dei soggetti interessati da questo provvedimento, che è riconducibile complessivamente, a oltre 182 soggetti, per un complesso di 400 annualità interessate. Molto più complesso è, però, determinare una previsione delle somme che saranno oggetto di questa restituzione, perché ciò sarà il risultato delle procedure di riscontro e di iscrizione a ruolo delle dichiarazioni dei soggetti interessati; particolarmente, bisognerà verificare quale ambito di applicabilità potrà avere la regolamentazione del *de minimis* per una più appropriata valutazione dell'effettivo ammontare degli aiuti che vengono così recuperati. Nel lavoro della Commissione, per il quale ringrazio i Presidenti, i colleghi delle Commissioni, il collega relatore Sinisi e i rappresentanti del Governo, si è introdotto anche un significativo emendamento teso a precisare che l'Agenzia delle entrate deve provvedere al recupero degli aiuti solo nell'effettiva misura di cui gli stessi sono stati usufruiti dalle società beneficiarie, ferma restando

In particolare, il comma 1 abroga l'articolo 2450 del codice civile, recependo così l'indicazione della Commissione europea che aveva avviato una procedura d'infrazione, mettendo in mora l'Italia per violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato della Comunità europea sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali. Come si legge nella relazione illustrativa del Governo, l'articolo 2450 del codice civile risulta attualmente privo di concreta attuazione nel sistema societario e, per di più, a fronte di tale sostanziale inutilità, esso appare in palese contrasto con la normativa comunitaria, caratterizzato com'è dall'attribuzione a soggetti pubblici della possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neppure soci; pertanto, se ne prevede l'abrogazione. I commi 2 e 3 sono finalizzati a recepire le indicazioni fornite dalla Commissione europea in merito alla corretta trasposizione della direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi, la cosiddetta direttiva sugli interessi e le *royalties*, che il Governo italiano aveva a suo tempo, nel 2005, recepito; è stata avviata però una procedura di infrazione, in quanto si è giudicato che la scelta operata con il decreto legislativo n. 143 del 2005 avesse ridotto l'ambito applicativo delle norme comunitarie e fosse sproporzionata rispetto alla finalità di prevenire eventuali abusi. Di conseguenza, le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo si uniformano a quelle prescrizioni e disciplinano le modalità di recupero anche tramite la previsione della compensazione delle ritenute così restituite. Anche in questo caso, si è lavorato a definire ulteriormente riferimenti al comma 4 in cui si stabiliscono i compiti assegnati all'Agenzia delle entrate, che devono essere svolti con risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente, quindi senza maggiori oneri. Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, che sono stimati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provveda con una parte delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all'articolo 1, da far affluire in un'apposita contabilità speciale intestata al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. finanze. Anche in questo caso, attraverso il lavoro in Commissione si è introdotto nel provvedimento, con la modifica dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, un adeguamento della legislazione interna alle numerose pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee in tema di tasse di concessione governativa sulle società. Ci si riferisce, in particolare, alle diverse pronunce di illegittimità dei tributi previsti per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, i quali non abbiano carattere remunerativo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo d'interesse generale quale è quello della pubblicità degli atti sociali.

ed abroga la disposizione che prevedeva l'inapplicabilità dei divieti di sponsorizzazione di eventi o attività quando questi si svolgevano esclusivamente nel territorio dello Stato. Secondo la relazione governativa, l'abrogazione di tale norma si è resa necessaria per dare immediata risposta ai rilievi formalizzati dalla Commissione europea, dapprima con una procedura di infrazione e quindi con ricorso alla Corte di giustizia. Nel ricorso la Commissione europea sostiene che la legislazione italiana introduce una deroga al divieto di sponsorizzazione non prevista dalla direttiva, che vieta appunto la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri. In proposito, desidero ricordare, ed informare l'Aula, che attraverso la discussione che si è svolta in Commissione si è definito un importante ordine del giorno, del giorno, proposto in Commissione e che il Governo ha dichiarato di accogliere, che dà mandato proprio al Governo di precisare quali possono essere i profili di attività di promozione e di sostegno da parte di *sponsor* che non rientrino e non ricadano nella logica e nel principio degli effetti transfrontalieri. Questo per la possibilità che vi siano destinazioni di somme utili ad interventi che privilegino e di cui possano beneficiare le comunità locali e i territori, per interventi di riqualificazione, di recupero e di sostegno ad attività di salvaguardia e tutela di tradizioni, beni culturali e quant'altro. Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, per la parte di cui sono chiamato a fare la relazione, richiamo, per gli articoli introdotti attraverso il lavoro in Commissione, la particolare rilevanza dell'articolo 5-*bis*, che introduce norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro. Anche in questo caso le norme che qui sono proposte alla valutazione ed al voto dell'Assemblea sono tese a porre rimedio all'incompatibilità della normativa italiana concernente i consulenti del lavoro con i principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e di libero stabilimento all'interno della Comunità e ad evitare quindi la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia. Infine, come

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il completamento della relazione del collega Barbolini sarà molto breve, per quanto mi concerne. L'articolo 2, che non è stato trattato, prevede sostanzialmente la messa a disposizione delle somme necessarie per promuovere la candidatura della città di Milano all'esposizione universale del 2015. L'articolo 4, nei commi che non sono stati trattati, concerne, in particolare al comma 2, le reti di telecomunicazione. vi era una procedura d'infrazione perché il nostro Paese, con le parole aggiuntive all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha posto dei costi aggiuntivi al diritto di accesso. Detta procedura d'infrazione, sarebbe sanata con l'abolizione delle parole di cui al comma 2. Al comma 3, invece, l'abrogazione è propedeutica a superare gli impedimenti che le società che producono, trasportano e vendono energia possano accedere ai servizi cosiddetti post-contatore. Il comma 4, infine, concerne il diritto d'autore per allineare il nostro Paese alle disposizioni vigenti nell'Unione Europea. L'articolo 5, signor Presidente, onorevoli colleghi, concerne l'immigrazione e si divideva, originariamente nel decreto, in due parti: la prima parte riguarda i permessi di soggiorno brevi, per visite, affari, turismo e studio, la seconda parte concerne la possibilità per le imprese comunitarie di assumere e di trasferire in qualsiasi parte dell'Unione Europea, personale anche se extracomunitario affidando la legittimazione soltanto alla dichiarazione e non al permesso di soggiorno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i lavori in Commissione sono proceduti i lavori in Commissione sono proceduti speditamente sulla base di un metodo che ha consentito di lavorare davvero all'unisono con tutti Gruppi politici e su tutte le proposte presentate dai singoli parlamentari. In particolare, voglio ricordare due punti sui quali abbiamo trovato una larghissima convergenza: i servizi post-contatore sono stati oggetto di un emendamento proposto da Rifondazione Comunista,

a seguito dell'approvazione in Commissione, su parere favorevole del Governo, di una questione che era stata già affrontata in sede di finanziaria e che viene comunemente denominata CIP6. Mi auguro che il lavoro di convergenza che è stato fatto in Commissione non sia pregiudicato da questa vicenda assai particolare e assai singolare e mi auguro altresì che si possa trovare una soluzione in Aula che renda spediti i nostri lavori e possa contribuire a ricostruire quel clima di collaborazione che in Commissione c'è stato durante il corso di tutti i lavori. Alla luce di tutto

il fatto che la stessa Commissione, e - spero - anche il Governo, voglia riesaminare, attraverso una sospensione, l'inserimento

a problemi che ci derivano da obblighi comunitari internazionali, ha bisogno della sua approvazione, anche perché ogni giorno di ritardo comporta, tra l'altro, oltre che inadempimenti, anche dei costi. il Governo presta particolare attenzione all'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento. È questa la ragione per cui durante i lavori della Commissione, in particolare sull'articolo 5, il Governo ha collaborato con i relatori, con il Presidente e con i membri della Commissione per risolvere nel modo migliore i problemi così da consentire a tutti

una parte è rimasta nel testo e un'altra è diventata un autonomo disegno di legge che la Commissione affari costituzionali ha già cominciato a discutere.

nel testo dell'emendamento, su cui i relatori e il Governo hanno dato parere favorevole e che la Commissione ha poi approvato. Al riguardo vi è un parere critico, negativo;

al punto tale che per questo potrebbe esservi un capovolgimento di quel clima che, invece, risolvendo i problemi relativi all'articolo 5, ci ha consentito di procedere positivamente durante i lavori della Commissione.

Mi auguro quindi che l'opposizione, apprezzando l'atteggiamento del Governo che, pur ribadendo un'opinione, riconosce la validità di un concorso parlamentare a più voci per arrivare ad una soluzione positiva del problema, da questo stesso atteggiamento tragga le conseguenze necessarie, ritirando quegli emendamenti che hanno - lo dico per brevità - carattere ostruzionistico, in modo tale da consentirci di procedere all'approvazione definitiva del provvedimento.

intervengo anch'io per apprezzare la decisione del Governo e dei relatori di ritirare l'emendamento 4.0.100.

di attuazione di obblighi comunitari, di infrazioni, di sentenze della Corte di giustizia e di procedure che contestano all'Italia inadempimenti, si registra un vasto consenso sul quale, qualche volta, manca una punta di criticità. Occorrerebbe valutare in maniera più approfondita il contenuto dei rilievi comunitari prima di arrivare a un provvedimento

da registrare nella procedura della legge comunitaria annuale, perché appare strano che ci si trovi di fronte

Ho seguito il dibattito sulla legislazione comunitaria svoltosi in quest'Aula; non so se bisognerà votare un documento - immagino di sì - però credo che occorra compiere una riflessione su tali procedure e verificare se il ritardo sia dovuto a inghippi e questioni di carattere legislativo interno, oppure se piuttosto non sia dovuto agli uffici o allo scarso coordinamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea. tra l'altro, solleva contestazioni di infrazioni comunitarie e alcune di queste norme mirano proprio a riparare a tali procedure, ma non è detto che la Commissione europea abbia sempre ragione. Quindi, occorrerebbe anche valutare meglio se la Commissione europea, nell'iniziare queste procedure e nel contestare questi fatti, trovi un fondamento valido alle proprie obiezioni. Il primo problema posto da questo decreto-legge

è in ritardo nell'attuazione della normativa comunitaria, pur avendo sostenuto degli sforzi notevoli. Anche l'ultima legge comunitaria contiene decine e decine di direttive per le quali è disposta

carico di valorizzare al massimo il principio di sussidiarietà ma anche di intervenire in materia di fonti legislative, prevedendo che alcune leggi particolari di origine comunitaria avessero vigenza immediata nell'ordinamento giuridico interno. Questo oggi non è e finché non avverrà, ferma restando la riserva per questa ipertrofia legislativa comunitaria, saremo sempre di fronte a ritardi nell'attuazione delle direttive. Fatta questa affermazione di metodo, voglio anche dare atto della

Anche da questa valutazione nasce la disponibilità di tutta la Commissione, come immagino di questa Aula, per evitare che questo provvedimento,

Purtroppo, il Governo ha usato lo strumento improprio del decreto-legge per intervenire su una materia

ma meno incidente rispetto al necessario. Da ciò derivano una serie di problemi sia di ordine politico che di ordine procedurale. Rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, relativo a materia comunitaria e a infrazioni che sono state richiamate, abbiamo assistito al tentativo da parte di settori della maggioranza di introdurre norme estranee. Le norme estranee erano anche quelle relative al cosiddetto finanziamento all'energia da fonti rinnovabili. In Commissione abbiamo ripetuto più volte, in maniera anche decisa, che era necessario seguire un percorso diverso, di non introdurre cioè quella norma un decreto-legge. Tra l'altro va ricordato come lo stesso Governo il 22 febbraio

stato tagliato fuori da tutto il dibattito. Allora l'UDC ha svolto una opposizione costruttiva, tesa al miglioramento del testo su alcuni punti nodali del decreto. Mi riferisco, in particolare, alla questione del *post* contatore; la soluzione che è stata individuata attraverso un confronto costruttivo ci soddisfa perché la questione presentava molto inesattezze all'origine. La questione non è di poco conto e ci riporta al complesso problema delle municipalizzate. La questione delle municipalizzate è il cuore delle questioni che abbiamo noi di fronte e che dovrebbero far riflettere rispetto alle scelte che stiamo per fare. E' in un certo senso collegata anche alla disciplina dei servizi pubblici locali, sulla quale dobbiamo fare una operazione verità. Toccare i servizi pubblici locali significa toccare un potere mostruoso, sia in termini di PIL, sia politici, sia di occupazione. Per chiudere la procedura di infrazione fu introdotto l'articolo 35 della legge finanziaria 2001, poi abrogato. In Italia vi è il cosiddetto nanismo delle microimprese; in Europa invece vi sono grandi imprese come la RVE che copre tutte le imprese italiane messe insieme: è grande 10 volte l'ACEA, la AEM di Milano, la AMGA di Genova, la HERA di Bologna, la ASM di Brescia. La preoccupazione allora era quella di non mettere in gara tutto, se non si intendeva mettere a rischio la struttura italiana a svantaggio dei consumatori e delle imprese. Quella era la prima questione. Rientrano nei servizi pubblici locali che devono garantire universalità del servizio, cioè raggiungere anche gli utenti non economicamente convenienti, dove non vi è dunque convenienza all'investimento se non nel lungo periodo. La colonizzazione straniera avrebbe determinato conseguenze possibili negative sopratutto sui consumatori italiani, tenendo tariffe più convenienti nei Paesi d'origine ed invece remunerandosi nel nostro mercato a svantaggio dei nostri utenti. Il mercato è competitivo se esistono i *competitor* e non i monopoli. Oggi in Italia ed ancor più nel 2003 non esistevano e non esistono soggetti privati con forze sufficienti a competere a livello nazionale ed europeo. ed europeo. Gli unici competitori sono quelli pubblici. A ciò va aggiunto che un altro problema è derivato dal novellato Titolo V della Costituzione che attribuisce - non citandola - la materia residuale alle Regioni in via esclusiva, all'*ex* articolo 117, come affermato dalla sentenza della Corte n. 272 del 27 luglio 2004. Unica competenza rimasta allo Stato è la tutela della concorrenza, che delinea l'ambito entro il quale muoversi. La concorrenza vuol dire come affidare la gestione del servizio riportando nella legittimità comunitaria la normativa precedente, che era oggetto di procedura di infrazione comunitaria dal 1999. E la riforma ha individuato tre modalità di intervento perfettamente congrue al diritto comunitario, che, se correttamente applicate e stimolate con le normative di settore e di competenza regionale, avrebbero portato al risultato di stimolare la crescita mediante aggregazione degli operatori nazionali, senza rischi di una gara comunitaria che li avrebbe visti soccombenti. Questo appunto attraverso la famosa lettera *c)*, cioè l'affidamento corretto*in house* senza gara. Successivamente, si sarebbe dovuto stimolare l'apertura ai privati anche alle società, mediante l'applicazione corretta della lettera *b)*, cioè partenariato pubblico-privato, per poi passare con tranquillità alle gare. Questi tre principi dovevano trovare concreta ed effettiva applicazione entro il regime transitorio del 31 dicembre 2006, concordato esplicitamente con la Commissione europea. A quella data tutti gli affidamenti non conformi a queste modalità di affidamento sono decaduti, come espressamente stabilito dall'articolo 115, comma 15, del Testo unico degli enti locali. La riforma La riforma proposta, facendo finta di richiamarsi alle liberalizzazioni del settore pubblico degli enti locali, ma in realtà leggendo congiuntamente il testo Lanzillotta e gli emendamenti del Governo, ha come unico scopo quello di cancellare la data del 31 dicembre 2006 appena scaduta, prevedendo un ulteriore regime transitorio fino alla data del 2011, alla quale tutti gli affidamenti, compresi quelli illegittimi, rimarrebbero in piedi. Ciò fa saltare l'accordo con l'Unione Europea. Quindi, il testo proposto dal Governo stravolge completamente gli accordi italiani con la Commissione europea, pertanto ci si chiede se questo Governo abbia agito contro il precedente Governo, che aveva concordato le linee della riforma con l'Unione Europea. Proprio la vicenda delle liberalizzazioni Presidente, devo indurci a qualche riflessione. Assistiamo a questa coop partito-azienda, con giganteschi intrecci d'interessi economici‑politici conflitti di interesse (gli stessi uomini che hanno un ruolo dirigente nelle società e anche nei partiti). Vediamo l'affermazione di un cosiddetto capitalismo regionale, in luogo del capitalismo di Stato. Nel caso, ad esempio, della HERA abbiamo una società con 45 miliardi di fatturato, più del 3 per cento del PIL, migliaia di dipendenti, 7 milioni di soci, 12.500 cooperative aderenti. Dove è lo scandalo? Nella mancanza di trasparenza, di *accountability*, nella disparità di trattamento rispetto alle società di capitali, soprattutto nella tassazione, che consente la deducibilità del 70 per cento dell'IRES dalla base imponibile, dalla deducibilità integrale degli utili destinati a riserve obbligatorie, la cosiddetta riserva legale a fondi mutualistici, deducibilità del 70 per cento degli utili destinati a riserva volontaria, purché indivisibili. A ciò va aggiunta la facilitazione dei prestiti sociali al 12,50 per cento, anziché al 27 Quindi, stiamo parlando di una *multi-unity* modello capitalismo rosso, dove anche recentemente il Governo Prodi ha inserito la

La HERA serve 196 Comuni dell'Emilia-Romagna su 341, con un bacino di utenza di 2,5 milioni di abitanti, che ha registrato 59 milioni di utili nel primo semestre 2006, che punta ad allearsi con AEM Torino e AMGA di Genova,

cui non interessano i problemi del territorio e la qualità dei servizi, aumenta le tariffe, non fa investimenti, sfrutta e licenzia i dipendenti, mentre il *management* è costituito da una schiera di privilegiati che pensano solo al successo personale. Queste sono le affermazioni di qualcuno che evidentemente conosce bene le cose. Se guardiamo la tariffa dell'acqua,

ha espunto l'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali» nel famoso emendamento, ribaltando l'obiettivo del provvedimento: distorsione della concorrenza, alterazione del mercato e parità tra gli operatori. Bersani, invece di liberalizzare - vogliamo fare un'operazione verità - difende i monopoli costituiti dalle municipalizzate con le Coop come azionisti. Presidente, mi avvio alla conclusione, abbiamo fatto una grande battaglia per difendere il post contatore, che comporta la difesa delle piccole e medie imprese e degli artigiani. La soluzione che è stata adottata ci convince, nel senso che abbiamo determinato le condizioni affinché non ci siano situazioni di monopolio, ma ci sia una reale concorrenza, né una separazione delle società che avrebbe alterato la concorrenza nel nostro Paese. Per queste ragioni, siamo soddisfatti delle soluzioni adottate, perché dietro quell'operazione c'era - per così dire - una difficoltà per migliaia di persone, di aziende, di famiglie, migliaia di occupati. Abbiamo inteso tutelare i piccoli rispetto ai grandi. Abbiamo anche cancellato quella furbata che si voleva introdurre attraverso l'emendamento concernente i CIP6; riteniamo corretto utilizzare il disegno di legge 1347, appunto la soluzione che il Governo ha individuato, attraverso un percorso a parte. Quindi, evitiamo di utilizzare decreti-legge per realizzare operazioni che servono soltanto a salvaguardare pezzi di questa maggioranza che si trova in difficoltà, che non riesce a trovare una sua coesione e quindi penalizza gli interessi del Paese.

Anche in questa occasione il lavoro dell'opposizione ha consentito di evitare un danno grave al Paese, attraverso l'introduzione surrettizia in questo decreto-legge di una norma che escludeva il contributo CIP6 alle fonti assimilate alle rinnovabili, come la frazione non biodegradabile dei rifiuti. In particolare, tanto per essere chiari, quella disposizione andava a porre un freno allo sviluppo dei termovalorizzatori nel nostro Paese. L'opposizione ha fatto fino in fondo il proprio dovere, ha sventato questa iniziativa, che era stata sbandierata dalla sinistra massimalista come un grande risultato; per fortuna, con le nostre capacità, siamo riusciti ad evitare questo danno grave al Paese. Quindi, se oggi potremo dare il via libera a questo decreto-legge con un intervento parlamentare non contrastato, è evidentemente un risultato positivo da ascrivere all'iniziativa dell'opposizione all'interno di questo Senato. Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, non possiamo che sostanzialmente condividerne le finalità, anche se non possiamo negare che lo strumento che è stato adottato, un decreto-legge, a poca distanza di tempo dal varo della legge comunitaria,

provvedimenti di attuazione delle direttive europee devono essere varati, ciò deve avvenire mediante lo strumento proprio che è, appunto, la legge comunitaria. Per quanto riguarda i contenuti in generale del

le *lobbies* delle ex municipalizzate, da colossi che possono stritolare soprattutto gli artigiani ed i piccoli imprenditori. La soluzione che è stata individuata nel testo che oggi ci accingiamo a varare, con un emendamento fatto proprio dalla Commissione, è a soluzione equilibrata, che tutela e che garantisce i piccoli imprenditori, le piccole aziende, di fronte al tentativo che anche in questo caso era stato operato di comprimere gli spazi di libertà economica che sono loro riconosciuti. *(Applausi dal Gruppo*

un disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante alcune disposizioni volte ad attuare obblighi comunitari ed internazionali. Il provvedimento è stato definito una minicomunitaria, e in effetti è una minicomunitaria, anche molto mini da questo punto di vista:

è contenzioso aperto da parte della Comunità europea, della Commissione europea, o addirittura procedure di infrazione in corso o pronunciamenti di incompatibilità della nostra normativa con direttive europee sono in una quantità notevole. Mi auguro che con la comunitaria in corso di definizione si possa coprire l'insieme di tali materie su cui c'è un'esposizione che non mette in difficoltà soltanto dal punto di vista politico, cosa che pure conta nei rapporti con la Comunità europea, ma anche perché le infrazioni si pagano, per cui c'è un costo che l'Italia sta sopportando per il mancato adempimento ed il mancato adeguamento delle normative rispetto ai pronunciamenti o alle direttive dell'Unione europea. Pur tuttavia, queste prime materie sono importanti. Noi abbiamo lavorato nelle Commissioni riunite in maniera produttiva, pensiamo in questo modo di aver abbassato in qualche misura la quantità, se non altro, del contenzioso con la Comunità Europea e ci auguriamo che su questo terreno si faccia un lavoro,

all'insorgere di problemi sociali rilevanti: penso, una per tutte, alla questione delle quote latte, ma penso anche a tutta la normativa sull'ambiente e sulla tutela della fauna selvatica, dove l'Italia è praticamente inadempiente. Si è ritenuto (e da questo punto di vista l'intervento del Governo stamattina è stato apprezzabile per la chiarezza e per la lealtà anche se da parte mia non condivisibile in pieno nel merito e nel contenuto) di limitare il campo degli interventi modificativi di questo disegno di legge non includendo altri elementi, altri elementi, quali potevano essere appunto quelli legati al finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili. Dato che

che sarebbe dovuta diventare parte del maxiemendamento e che invece nel maxiemendamento è stata letteralmente stravolta, anzi capovolta nel suo

che il Governo ha provveduto, come si era impegnato a fare, a presentare un disegno di legge in materia. Tale disegno di legge è già al Senato e stamattina

consente di utilizzare i soldi, i finanziamenti che provengono dalle bollette dell'energia elettrica che ognuno di noi paga, e che paga in funzione del fatto che questi finanziamenti debbano servire a sviluppare le fonti alternative, non a produrre energia dai rifiuti o a finanziare la produzione di energia dai residui delle lavorazioni industriali nella raffinazione dei prodotti petrolchimici. Quindi, io penso che non ci sarebbe stato niente di strano, però, coerentemente e lealmente ci atteniamo ad un orientamento che la maggioranza e il Governo ci chiede aderiamo a questa procedura. Analogamente, abbiamo aderito alla procedura - anch'essa, devo dire la verità, discutibile relativa allo stralcio di gran parte dell'articolo cinque. Capisco che tra di noi in quest'Aula, al Senato esistano questioni politiche aperte

la legittima esigenza di ciascuno di noi e di ciascun Gruppo di segnalare la propria posizione e il proprio ruolo si fermasse alla soglia di quello che

non fa bene all'economia del Paese. Ciascuno di noi, in una o più sedute di Commissione e d'Aula, può segnare un punto a proprio vantaggio in una sorta di battaglia navale, ma

che vogliono venire in Italia per motivi di studio, di turismo, di lavoro, di prestazione professionale, di impegno universitario o per attività economiche

che, a fronte di un pronunciamento della Corte di giustizia europea, sia stata trovata una soluzione di grande equilibrio e buon senso sulla questione dei servizi «post-contatore»

in maniera arbitraria alle imprese distributrici e detentrici delle reti, e quindi distributrici del del gas e dell'energia elettrica, di intervenire nei servizi interni, nei servizi dentro il domicilio, oltre il collegamento oltre il collegamento ai contatori, però la soluzione proposta nel decreto avrebbe fatto sì che si sarebbe

capace di mettere fuori mercato una miriade di imprese piccole e medie e soprattutto di imprese artigiane che sono quelle che operano a domicilio nei servizi di installazione e manutenzione

nella discussione in Commissione i consensi e la possibilità di ulteriore affinamento ha reso possibile su questa materia un equilibrio tra

Non voglio soffermarmi sul fatto che questioni di questa natura, cioè l'esercizio delle attività di servizio privato, sono state alla base di una discussione enorme che si è sviluppata perfino

aver trovato un punto di equilibrio tra il ruolo e l'interesse delle grandi imprese di distribuzione dei servizi a rete e la salvaguardi del ruolo e dello spazio della piccola e media impresa e delle imprese artigiane, ritengo sia estremamente importante. Ci sono altre norme nel decreto che sono state aggiustate, elaborate, rielaborate, ridefinite; mi pare che quella relativa proprio al controllo delle materie dei prodotti chimici, a salvaguardia della salute individuale, ma anche della tutela ambientale, sia una norma molto utile al nostro Paese e molto impegnativa. Credo che, in sostanza, si sia fatto un buon lavoro. Se posso, solleciterei il Governo ad effettuare una ricognizione compiuta delle materie oggetto di procedura di infrazione comunitaria assoggettate a pronunciamenti della Corte o dell'Unione, in modo tale che davvero si possa rapidamente, con la legge comunitaria, sanare tutte insieme le partite che sono ancora oggetto di contenzioso. Questo eliminerebbe, anche nel confronto politico tra di noi, la reciproca accusa

Signor Presidente, inizio questo mio breve intervento rapportandomi e collegandomi all'intervento del collega Bonadonna, che, intervenendo prima di me, ha sostanzialmente giustificato questo provvedimento con l'esigenza di superare il contenzioso esistente con l'Unione Europea, creando quindi le condizioni per una normalizzazione del rapporto. Credo innanzitutto di dover dire, con grande franchezza, che, anche nei rapporti con l'Unione Europea (parlo da europeista), non bisogna tenere un atteggiamento soccombente e debole. Molte volte l'Unione Europea ha posto delle problematiche ed ha fornito degli indirizzi assolutamente irricevibili, quindi contestabili sul piano della dottrina e delle motivazioni.

nella realizzazione dei provvedimenti, perché quanto più i provvedimenti contenenti al proprio interno questioni relative a rapporti con l'Unione Europea vengono infarciti da norme che non hanno alcun titolo per stare all'interno dei provvedimenti medesimi, tanto più difficile sarà semplificare la materia. Quello di oggi è un esempio lampante di quanto sto dicendo in questo momento. Ho qui la tabella

ormai si parte da un assunto assolutamente sbagliato, quello della sostanziale equiparazione tra le direttive e i regolamenti, dimenticando che c'è una differenza di fondo sotto il profilo giuridico e una differenza sostanziale sotto il profilo normativo. Mentre per i regolamenti c'è l'obbligatorietà, da parte di uno Stato membro, a recepirli, tutto questo non avviene, né può avvenire, per le direttive. Le direttive hanno lo scopo precipuo di avvicinare ed armonizzare gli ordinamenti giuridici nazionali, ma non hanno l'obbligo di determinarli. Equiparare, dunque, una violenza, una contraddizione in termini, anche perché non possiamo uniformarci in maniera totale, altrimenti perderemmo quello spirito unitario della nostra storia che, invece, credo vada mantenuto all'interno di un contesto europeo. Fatta questa premessa, aggiungo che Alleanza Nazionale osserva, valuta e apprezza l'atteggiamento che il Governo ha ritenuto di assumere riguardo alle norme contestate.

cercando di costruire, non sul piano della mera opposizione, ma su quello di una sana e corretta dialettica interna, le condizioni per migliorare questo provvedimento e per evitare sostanzialmente che esso potesse procurare danni al Paese. perché al di là del merito - che non condividiamo - anche le due materie principali alle quale abbiamo fatto riferimento non dovrebbero mai poter essere oggetto di decreti-legge. dovrebbero costituire oggetto di dibattiti approfonditi all'interno del Parlamento attraverso lo strumento del disegno di legge che è l'unico in grado di garantire questa effettività.

costituisce oggi un bubbone che negli anni non siete riusciti a estirpare. Vi è bisogno, quindi, di un franco dibattito su questo tema e ciò non può avvenire con lo strumento del decreto-legge. Così come di un sano dibattito ci sarebbe bisogno riguardo al tema dell'immigrazione rispetto al quale al quale non possono porsi in essere iniziative contraddittorie: non si può, da un lato, intervenire con segmenti specifici all'interno di questo decreto-legge, dall'altro, anticipando - osserviamo quanto avvenuto nei giorni scorsi da parte del Governo - un disegno di legge che, per certi versi, potrebbe anche contrastare con i provvedimenti inseriti all'interno dell'articolo 5. Sono queste le questioni importanti sulle quali abbiamo condotto una battaglia politica che ha dato un certo risultato. Ma di questo - ripeto - va dato atto all'opposizione per averla condotta con grande correttezza, ma anche al Governo e alla maggioranza per aver risposto con grande senso di responsabilità.

la nostra soddisfazione per aver stoppato per certi versi l'articolo 5. Ci ripromettiamo di ritornare sull'argomento per affrontarlo veramente in termini molto chiari e complessivi. Siamo

ma non intendiamo farlo in questa occasione perché siamo perfettamente consapevoli che, quando si raggiunge un risultato, non si deve lasciare spazio a nessuna polemica. polemica. Un altro principio importante che l'emendamento conteneva è quello della dissacrazione dei cosiddetti diritti acquisiti. Lo diciamo adesso non per fare polemica, ma perché anche per domani si possano creare le condizioni per evitare situazioni di questo genere, che imbarazzano molto e che a noi - lo debbo dire con grande senso di responsabilità - potrebbero addirittura far comodo perché ci sarebbe materiale per fare polemica politica in chissà quale maniera. Non vogliamo farla, però diciamo che abbiamo la necessità, di fronte ad un imponente corpo normativo, di uscire fuori con grande chiarezza su alcuni princìpi perché altrimenti non riusciamo ad ottenere i i risultati generali cui ho fatto riferimento precedentemente. Abbiamo determinato condizioni importanti per la tutela del cosiddetto post-contatore. Chi mi ha preceduto dai banchi dell'opposizione ha rappresentato una situazione reale che sicuramente ha l'attenzione dell'intero Paese. Noi, in un processo di deindustrializzazione che ha interessato l'Italia, non possiamo non assolvere a due princìpi: primo luogo, occorre tutelare il sistema delle piccole e medie imprese rispetto al quale è collegata la struttura portante dell'intero Paese, ma poi bisogna anche che da parte nostra si creino altre condizioni importanti, oltre

gli oligopoli, che diventano veramente il momento dell'affossamento delle regole della concorrenza interna ed internazionale. Oggi, purtroppo debbo dire che in Italia ancora qualche oligopolio, che esercita funzioni pesantissime e negative, sicuramente c'è. Siamo soddisfatti per il contributo che abbiamo dato; siamo pure soddisfatti per le risposte che abbiamo ricevuto; siamo soddisfatti certo come partito, ma lo siamo sotto ma lo siamo sotto il profilo politico ed istituzionale per il messaggio importante che abbiamo dato all'intero sistema Paese rispetto ad un insieme di regole che da oggi in avanti devono essere sicuramente rispettate. *(Applausi dal Gruppo* *AN)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà. Signor Presidente, questo decreto‑legge reca, come è stato detto dai relatori, dal Governo e dai colleghi che mi hanno preceduto, disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. In buona sostanza, questi obblighi discendono da due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: la prima attiene a delle risorse che si sarebbero dovute pagare e che non sono state pagate; l'altra, quella di cui all'articolo 3 del decreto, attiene a delle risorse che non si sarebbero dovute pagare e che invece sono state pagate. La soluzione - dice il Governo - è necessaria rapida, ma noi riteniamo che non sia altrettanto indolore perché la diversità per l'esecuzione delle due sentenze è specifica. Con riguardo all'articolo 1, le somme che in esecuzione della sentenza rivengono all'amministrazione dello Stato sono di quantificazione difficoltosa e non specificatamente rispondenti alle disposizioni della legge di contabilità, ma - guarda caso - hanno la stessa valutazione delle risorse necessarie, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, per coprire le necessità finanziarie di cui all'articolo 3, per l'esecuzione della sentenza che riguarda l'articolo stesso. Siamo cioè dell'idea che in questo caso si è voluta piegare l'inflessibilità della matematica, che deve stare a supporto della contabilità finanziaria e della contabilità dello Stato, alla logica del Governo; riteniamo cioè che il Governo abbia voluto arrogarsi il diritto di decidere sulla questione sé la matematica sia o no un'opinione, decidendo positivamente in tal senso; mentre noi riteniamo che sia doveroso da parte del Parlamento non essere altrettanto arroganti, così come ha fatto il Governo, e non siamo della stessa opinione rispetto alle necessità della legge di contabilità e alla necessità che la matematica, a supporto della legge di contabilità, abbia una sua

relazione tecnica abbastanza lacunosa. Questa infatti fa riferimento agli F24 successivi al periodo di riferimento, in quanto - dice il Governo - non è possibile risalire all'anno di imposta 1999 per quanto al titolo IRPEG, e fa una valutazione relativa al periodo 2001‑2004, non tenendo conto che nello stesso periodo, all'interno delle municipalizzate, è stato possibile che entrassero anche iniziative di tipo privato e che quindi le rivenienze, che vengono prese a base per la quantificazione, è ben possibile non siano quelle ipotizzate da parte del Governo in una possibile successione lineare di contribuzione. Questo significa le risorse rivenienti dall'articolo 1 sono forzatamente quantificate e - guarda caso - sono quantificate per quelle che successivamente sono indicate come necessarie all'articolo 3. Tuttavia, il fatto che ci fa supporre che tutto sia claudicante è che, mentre per l'articolo 3 non esisteva già una legislazione in materia, per quanto riguarda l'articolo 1 è lo stesso Governo che, nella relazione di accompagnamento del decreto, dice che già era operante una successioni di leggi e già era operante una legge specifica (la n. 266 del 2005), la quale aveva già dato possibilità al Ministero dell'interno di operare mediante un regolamento di attuazione. Il Governo però dice che il regolamento in proposito, un regolamento che - badiamo bene - era già stato possibile adottare per una legge del 2005 e che quindi bastava soltanto sollecitare, aveva dei tempi non compatibili con la definizione della procedura di infrazione in corso per rendere possibile la copertura delle risorse per l'impatto di cui all'articolo 3, si tira dentro lo stesso decreto come necessaria una disposizione per una infrazione per la quale già esisteva una disposizione vigente. A A questo punto, è ben evidente che si è voluto tirare dentro allo schema di copertura una copertura della quale non c'era assolutamente bisogno. Soprattutto, in Commissione, ci siamo espressi contrariamente, e continuiamo a essere contrari, che le risorse rivenienti dall'articolo 1 sono risorse di cui dovranno fare a meno gli enti locali; il Governo

sarà necessario sicuramente un maggiore «tiraggio» degli enti locali nei confronti dell'amministrazione dello Stato per queste minori risorse di cui avranno disponibilità. Sarebbe stato più opportuno disporre un blocco delle risorse nel capitolo di bilancio attinente agli enti locali sino a quando fosse stato appurato che la maggiore efficienza, richiesta dalla sentenza della Corte di giustizia europea, avrebbe determinato nell'amministrazione degli enti locali una rivenienza di risorse tali da poter pagare quanto chiestoci. Invece cosa si fa?

nella buona sostanza scoperta perché gli enti locali finiranno per richiedere le stesse risorse. Per tali ragioni, noi siamo assolutamente e completamente contrari alle modalità di copertura e riteniamo - lo ripetiamo ancora - che in questo caso il Governo stia

Signor Presidente, colleghi,

sono di rilevanza costituzionale. Pertanto, è evidente che anche l'obbligo di ottemperare agli impegni assunti nei tempi richiesti dal legislatore comunitario per gli Accordi internazionali per noi, come per tutti gli altri Paesi, adempimenti notevoli. Vorrei poi sollevare due questioni. In primo luogo, condivido l'eccezionalità dell'uso del decreto-legge,

Noi ci troviamo in una situazione di urgenza per due ordini di motivi: il primo è che nel 2006 abbiamo avuto un'interruzione della legislatura per la campagna elettorale, e quindi una serie di adempimenti ha subito dei ritardi. Il secondo è che - come i colleghi sanno - la stessa legge comunitaria, con le procedure previste, non è in grado, a causa della lentezza dei tempi di recepimento delle deleghe, di risolvere questioni di messa in mora e di infrazione come quelle che esame intende affrontare. In secondo luogo, forse giova ricordare che, in caso di mancata ottemperanza di una sentenza di inadempimento della Corte di giustizia,

Proprio l'Italia poi è parte in causa per l'alto numero di infrazioni pendenti. Come i colleghi forse sanno, la penalità di mora può oscillare tra un minimo di 11.000 euro e un massimo di 714.000 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo a partire dalla seconda sentenza della Corte. La sanzione forfetaria è di 9.920 euro; quindi, a partire dalla seconda sentenza della Corte si può applicare la sanzione forfetaria che è pari a circa 10.000 euro. Con le nuove disposizioni entrate in vigore a gennaio, si aggiunge una mora giornaliera che viene valutata di volta in volta, ma che ha una forbice da 12.000 a 714.000 euro al giorno. Per tali i colleghi vorranno apprezzare l'urgenza e l'utilizzo del decreto‑legge almeno per risolvere le infrazioni che sono in dirittura d'arrivo e che quindi non è interesse del Paese affrontare in questa sede.

il contributo che l'opposizione ha voluto dare, insieme con la maggioranza, per dare soluzione a una serie di questioni che ritenevamo urgenti e che speriamo di risolvere con il disegno di legge relativo relativo all'articolo 5. Mi pare però che, grazie alla collaborazione che si è manifestata, siamo in grado di risolvere almeno i problemi più urgenti, essendo inteso che la questione cui il Governo tiene molto, quella del CIP6, ha trovato un'altra sede per essere risolta.

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge in conversione, le parole "pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007". Il parere è altresì reso con i seguenti presupposti: - che la deroga prevista dall'articolo 2 del decreto-legge sia motivata da esigenze indifferibili connesse all'attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all'esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei principi in materia di affidamento posti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario; - che la contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge sia quella di cui all'articolo 27,

nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36,

e 1.0.20. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.20. Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 2.61 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel medesimo sia inserita una clausola di invarianza dei costi del seguente tenore: dopo la parola: "avvalendosi", inserire le seguenti: senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,". Sugli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80 esprime parere di nulla osta nel presupposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le deroghe in essi contenute siano motivate da esigenze indifferibili connesse all'attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all'esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei princìpi in materia di affidamento posti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario, analogamente a quanto già osservato sull'articolo 2 del testo. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1, (limitatamente al secondo periodo), 3.22, 3.23, 3.24, 3.0.500, 3.0.501 e 3.0.502. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.4. Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 3.31, nel presupposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il bilancio a legislazione vigente già sconti l'onere determinato dalla giurisprudenza comunitaria, recepito in prima istanza con atto amministrativo, risultando la modifica normativa un mero atto di adeguamento formale all'ordinamento comunitario. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2),

mentre il parere è di nulla osta sull'emendamento 5.0.1 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole: "Per gli anni 2008 e 2009", siano sostituite con le seguenti: "Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"; dopo la parola: "mediante", inserire la parola: "corrispondente"; dopo la parola "speciale," inserire le seguenti: "dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007," e sostituire la parola "apporre" con la seguente: "apportare". Esprime quindi parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

è relativo all'attuazione del Numero unico europeo di emergenza 112, che ha l'obiettivo principale di realizzare un sistema integrato, coordinato ed efficace per la gestione delle risposte alle chiamate di emergenza. Rispetto a questo obbligo comunitario,

il parere motivato di contestazione dell'infrazione, che per l'appunto porta il n. 2006/2114. Rispetto a questa materia

prevede di ripristinare le modalità già previste dal precedente Governo per la realizzazione del progetto, che si è servito all'epoca di due strutture di lavoro interministeriali, che hanno già rappresentato utilmente il Governo e che hanno già creato le condizioni, sia progettuali che di finanziamento, per la realizzazione del progetto. Il progetto prevedeva una fase iniziale di sperimentazione, che doveva realizzarsi sui territori delle Province di Salerno, Catanzaro e Palermo.

sarei disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, qualora dal banco delle Commissioni riunite venisse una richiesta di questo tipo. Si tratta di un provvedimento particolarmente delicato;

Governo:

intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico

Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, signori del Governo, il decreto-legge in oggetto poggia le proprie ragioni di necessità e urgenza su molteplici aspetti. È bene partire da qui per rispondere anche ad una serie di rilievi critici avanzati dall'opposizione, in primo luogo sull'opportunità, trattandosi di obblighi già scaduti, di riconoscere il potere al Governo di proporre provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti comunitari o a sentenze che comportino obblighi statali di allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. In secondo luogo, risulta quanto mai opportuna la necessità di rispondere adeguatamente, e con adeguata celerità, ad una serie nutrita di procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea all'indirizzo del nostro Paese su un ampio numero di aspetti normativi. Le Commissioni riunite sono state informate costituzione presso il Dipartimento per gli affari europei di uno specifico osservatorio sulle infrazioni comunitarie, al quale è stato affidato il compito di curare i rapporti con le varie amministrazioni nazionali coinvolte nel processo di adeguamento al diritto dell'Unione Europea.

attraverso l'esborso di salate multe europee, sia per altri due aspetti inerenti danni economici cui è esposto il nostro Paese. infatti, la nostra industria turistica vede deviati verso altre mete europee importanti flussi turistici provenienti da quelle classi abbienti che vanno emergendo dall'economia asiatica (senza dimenticare la protesta formale dell'ambasciatore giapponese in Italia perché i loro turisti non riescono ad arrivare agevolmente nel nostro Paese). Dall'altro, difficoltà emergono anche nei rapporti di lavoro che le nostre aziende di ogni dimensione

speriamo si possa risolvere nel modo più rapido il problema dei visti brevi per turisti, *manager*, professori e studenti che vengono a soggiornare nel nostro Paese, considerando il valore limitato e il carattere politicamente non molto rilevante delle disposizioni stralciate ed oggetto di infrazione comunitaria.

adeguatamente alle obiezioni sollevate più parti in Commissione, in particolare rispetto all'effettivo impatto della misura recata dall'articolo 4, dove l'evocazione del principio di libera concorrenza appariva debole e confusa in considerazione dell'obiettiva sostanziale posizione di vantaggio offerta alle grandi aziende operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas

all'esigenza di armonizzare pienamente l'ordinamento italiano con la direttiva comunitaria, anche se devo dire a me personalmente sono arrivate forti preoccupazioni, in particolare rispetto all'occupazione e alle prospettive per le quali l'introduzione e l'adeguamento di questa normativa comporterà dei problemi non solo di competitività ma anche di carattere occupazionale. Infine, prendo atto, anche se con rammarico, della decisione assunta in merito al cosiddetto emendamento CIP6 approvato in Commissione con il parere favorevole del Governo, già convenuto

di piena assunzione dei princìpi lì contenuti. Mi auguro che l'accordo raggiunto, che vede il consenso e l'impegno per un *iter* legislativo accelerato, trovi i dovuti e conseguenti comportamenti da parte di tutti. Vorrei solo ricordare quel proverbio che dice che il buongiorno si vede dal mattino; vorrei augurarmi, in questo caso, che tale proverbio venga ad essere smentito. Vorrei, infine, ricordare, a chi durante il dibattito ha polemizzato e sottolineato la sua contrarietà rispetto a questo emendamento, che non si tratta di pretese o ricatti di qualche piccolo Gruppo,

la preservazione del sistema in cui viviamo, che ha raggiunto livelli vicini al rischio del collasso. Con queste considerazioni, per questi e con il rammarico espresso rispetto a quest'ultimo punto, anticipo il voto favorevole del mio Gruppo, a nome del quale sono intervenuto.

Signor Presidente, colleghi senatori, con il decreto-legge al nostro esame il Governo, per fare fronte ad obblighi comunitari ed internazionali, è ricorso allo strumento normativo d'urgenza, con contenuti solo apparentemente eterogenei, ma resi unitari dal comune scopo di provvedere ad obblighi ed impegni di fonte sopranazionale. È stato puntualmente rilevato durante l'esame in Commissione che la legge comunitaria per il 2006 è stata approvata dal Parlamento con notevole ritardo e che l'introduzione di ulteriori emendamenti, volti a recepire direttive in scadenza, avrebbe comportato un'ulteriore dilazione nella conclusione dell'*iter*. Per queste ragioni, il Governo si è orientato ad adottare il decreto-legge, in luogo del ricorso alla Legge comunitaria, per consentire in tempi rapidi di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea: ciò eviterà l'irrogazione di multe assai gravose conseguenti alle condanne per infrazione. e l'urgenza del decreto, pertanto, si collegano in via generale agli obblighi sopranazionali di adeguamento del diritto interno, degli articoli 117 e 11 della Costituzione. Passando rapidamente al merito del provvedimento, mi sono battuto affinché una norma molto rilevante e delicata, attinente all'annosa questione della gestione dell'emergenza rifiuti, trovasse collocazione in una sede diversa rispetto alla conversione di un provvedimento urgente. Accolgo, pertanto, con estremo favore, la decisione saggia del Governo, condivisa dalla Commissione, seguita al mio suggerimento e a quello di altri, di stralciare l'emendamento 4.0.100, concernente una norma della legge finanziaria articolo l) che prevede incentivi e finanziamenti indispensabili per l'utilizzo dei termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti. Tale emendamento verrà trasformato in autonomo disegno di legge, che potrà essere adeguatamente discusso e approfondito. Altra norma cui vorrei fare rapidamente cenno è quella contenuta in una mia proposta emendativa, accolta come ordine del giorno dall'Assemblea, concernente l'attivazione del Numero Unico Europeo 112 per la gestione delle emergenze. L'Italia ha accumulato gravi ritardi per l'attuazione effettiva del progetto sul numero unico di emergenza, progetto per il quale il CIPE ha già stanziato 9, 7 milioni di euro e, pertanto, la Commissione europea ha avviato formalmente una procedura di infrazione. L'ordine del giorno indica termini certi per dare avvio alla fase di sperimentazione nelle tre province di Salerno, Catanzaro e Palermo e alla fase operativa del progetto su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2007.

esprimere solo poche considerazioni rispetto a quanto già detto in sede di discussione generale. Meritano - a mio avviso - di essere richiamate alcune questioni. In particolare,

Abbiamo difeso gli interessi dei più deboli rispetto alle posizioni dominanti nella distribuzione di energia

5, 2 miliardi di euro, che interessa 22 milioni di abitazioni, 121.000 imprese artigiane e 309.000 addetti. Queste sono le cifre messe in campo.

della mera abrogazione. Per queste ragioni, pur esprimendo soddisfazione per la soluzione adottata rispetto ad alcune questioni, preannuncio il voto di astensione del gruppo UDC sull'intero provvedimento.

e il rappresentante del Governo che hanno seguito in questa fase il lavoro di elaborazione e di definizione del disegno di legge.

Quando mi riferivo all'esigenza dell'Italia di raccordarsi e chiudere tutti i contenziosi con l'Unione Europea e con la Commissione,

troppo spesso e troppo colpevolmente i Governi del nostro Paese, spesso e volentieri, non hanno difeso le loro ragioni

un cammino virtuoso, invece che insistere in quello vizioso e peraltro viziato. Il CIP6 è uno dei punti di vizio. La Germania La Germania può prendere ed anzi è alla ricerca dei rifiuti della Campania perché i termovalorizzatori tedeschi non hanno più rifiuti solidi urbani tedeschi da bruciare, perché stanno attuando un'altra politica: una politica di riduzione dei rifiuti e di riciclaggio degli stessi. Non possiamo continuare su questa strada. Da questo punto di vista, voglio sottolineare il senso di responsabilità con cui abbiamo oggi accolto le valutazioni e il suggerimento del Governo. Vogliamo anche ribadire che l'impegno, assunto dal Governo

su cui - se leggete i giornali di oggi possiamo averne un'ulteriore conferma - le democrazie di questo nostro Continente hanno capito che ci sono elementi di valore, non soltanto civico e civile, ma anche economico e strutturale, che vanno salvaguardati. Da questo punto di vista, l'ambiente in cui si sviluppa la vita e l'attività umana è uno di questi.

vediamo che la buona volontà è prevalsa, così come la correttezza dei rapporti politici tra maggioranza e opposizione. Devo anche sottolineare la serenità con cui il Governo ha seguito il processo di formazione di questo provvedimento.

volte il buonsenso è l'unica via per cercare di fare politica in un Parlamento, in un'Aula, quale quella del Senato, con una maggioranza così risicata da parte del Governo e quindi della maggioranza dei partiti.

abbiamo fortemente contribuito alla definizione di alcune norme significative di questo provvedimento. Parlo, ovviamente, dell'articolo 5 e dell'articolo 4. All'articolo 4 c'era un emendamento soppressivo presentato dal senatore Valditara e da me: lo abbiamo ritirato perché abbiamo contribuito a definire una formulazione nell'articolo 4 che coniughi da una parte la necessità di rispettare gli orientamenti, le norme internazionali e dell'Unione Europea, quella di favorire la piccola e media industria del nostro Paese. Con la formula che è stata trovata da tutti noi pensiamo di aver dato una risposta, di aver aumentato le garanzie di concorrenza, di aver difeso anche in senso nazionale l'interesse dei piccoli

perché non affronta un tema che verrà affrontato nelle prossime scadenze parlamentari. È stato già preannunciato che ci sarà da parte del Governo una proposta per rivedere la Bossi-Fini; in quella sede sede ci confronteremo ma sarà una sede solo a ciò deputata, limitata a questo delicatissimo problema che riguarda proprio l'immigrazione e l'emigrazione. avvio alla conclusione di questo mio intervento facendo qualche osservazione: nemmeno questa volta abbiamo rinunciato, nella nostra responsabilità politica, a cercare di trovare punti di convergenza, senza inciuci, con un confronto leale e corretto, soprattutto quando si tratta di materie che riguardano la posizione dell'Italia in campo europeo e in campo internazionale. Certamente, avere da parte dell'Italia, correttezza di rapporti con l'Unione Europea, nei vincoli, nelle indicazioni e nelle direzioni, essendo anche un obbligo costituzionale previsto dall'articolo novellato 117 della Costituzione,

Sicuramente, gli amici della Camera hanno torto, però, non vi è dubbio che un maggiore rigore nella valutazione degli emendamenti, quando si tratta di decreti-legge,

l'occasione per ricordare a noi stessi quanto fosse lontano il tempo in cui alcune forze politiche, che - vivaddio - oggi sono tutte con noi europeiste, scrivevano nelle città d'Italia: Europa è uguale a fame. Come è ancora tanto lontana l'epoca in cui alcuni parlamentari, tra cui un mio maestro, andavano in giro, durante la campagna elettorale, per predicare l'Europa e per dire che essa era la riforma delle riforme. È stata oltremodo virtuosa la previsione di una legge annuale che impone al Parlamento una sorta di diario per recepire le direttive comunitarie, la cui

hanno snaturato la natura asettica - perché tale dovrebbe essere - di un provvedimento di politica internazionale, e segnatamente di politica comunitaria, qual è la legge comunitaria annuale. Allora, per esplicitare il nostro disappunto per questi tentativi, che se non fossero stati sufficientemente vanificati avrebbero fatto di questo un pessimo provvedimento, e perché ciò sia di monito

Signor Presidente, in primo luogo, mi corre l'obbligo di ringraziare il Governo per la disponibilità che ha dimostrato nella partecipazione attiva al confronto svoltosi nelle Commissioni 1ª e 6ª riunite. A tal proposito, vorrei ricordare la presenza ai nostri lavori dei ministri Rutelli e Bonino. Un giusto ringraziamento credo vada rivolto anche ai relatori e ai Presidenti delle Commissioni. Vorrei sottolineare, in termini positivi e in modo formale, il positivo confronto che si è realizzato su questo difficile provvedimento tra maggioranza e opposizione. Nel merito, va osservato, sicuramente in termini positivi, il modo in cui sono state affrontate le questioni proposte all'articolo 1 del provvedimento. Si tratta di un tema molto delicato e su questo si è cercato, nel rispetto delle prescrizioni date, di impostare procedure e modalità che tengano conto delle esigenze e delle prerogative dei Comuni e delle aziende, pur nei limiti consentiti. Da tale punto di vista, credo vada evidenziato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno. Inoltre, va osservato in termini positivi quanto previsto all'articolo 4 con riferimento alle attività post-contatore**,** perché credo si sia trovato un giusto equilibrio tra le necessità di ottemperare le prescrizioni comunitarie e, contemporaneamente, di corrispondere alle esigenze degli operatori, in particolare delle piccole e medie imprese artigiane. Infine, voglio segnalare l'adeguamento della nostra legislazione sul tema dell'attività dei consulenti del lavoro. Per tutti questi motivi, il Gruppo dell'Ulivo esprimerà un voto favorevole. Presidente, i Gruppi dell'opposizione hanno dichiarato un voto di astensione. Io ho argomentato poc'anzi la mia contrarietà, già espressa in Commissione bilancio, per

**Il Senato approva.**

avendo concluso anticipatamente i nostri lavori, alle ore 13, è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Noi torneremo a riunirci alle ore 16,30

a Serre, in provincia di Salerno, decine di cittadini, rappresentanti di comitati ed amministratori locali che presidiavano l'oasi di Persano, per impedire l'inizio dei lavori di una discarica decisa dal commissario Bertolaso. Non voglio entrare nel merito,

di sintesi e anche di mediazione e mentre un decreto sostiene che ogni decisione va presa d'intesa con gli enti locali,

delle cariche che hanno coinvolto il sindaco di Serre, alcuni assessori, il Presidente dell'Ente Parco e, soprattutto, cittadini. Ebbene, come volete che le popolazioni possano credere alla politica se, in queste ore, non sappiamo se la delegazione dei sindaci verrà tra un'ora, perchè nessuno si vorrà muovere se non ha la certezza che vi è la garanzia di alcune regole? Chiedo, Presidente, un suo intervento a tutela del ruolo di sintesi e di sindacato ispettivo del Senato e delle sue Commissioni. Agenzie di stampa spagnole - la principale è la EFE - riferiscono che, sin da lunedì scorso, truppe italiane e spagnole stanno conducendo un'offensiva militare contro i talibani, la più rilevante dall'inizio di quest'anno. Questa offensiva è sotto il comando del generale italiano Antonio Satta, ma la cosa più grave per cui ho chiesto la parola è che il Ministero della difesa italiano smentisce, mentre il Ministero della difesa spagnolo conferma. Ora, ci troviamo in una situazione di estrema delicatezza, tra l'altro siamo alla vigilia del voto che il Senato deve dare sul rifinanziamento della missione, ed è estremamente grave che il Ministro della difesa, in modo molto imbarazzato - posso leggere testualmente dica che le truppe italiane non sono impegnate, quando proprio gli spagnoli ci comunicano che il comando è sotto la direzione del generale italiano Satta. Signor Presidente, sarebbe urgentissimo in questa situazione che il Governo venisse a riferire in Senato e che dicesse la verità, soprattutto nel momento in cui un alleato come il Governo spagnolo non lo segue nella smentita, anzi, e che le agenzie di stampa spagnole non sono state smentite da alcuno.

e, immediatamente dopo, vi è stata l'immissione in commercio di detto farmaco. È un fatto gravissimo perché, durante quell'audizione, era stato detto che ciò sarebbe avvenuto dopo un certo periodo di tempo. si è determinato anche un pericoloso conflitto di interesse rispetto alle posizioni che coincidevano su questo farmaco. La inviterei, a sollecitare il Governo a dare una risposta su questo problema che ha suscitato vivissimo allarme nell'opinione pubblica ed anche nello stesso Parlamento. Una seconda questione

responsabilità del Ministro delle finanze *pro tempore* in relazione al provvedimento con il quale era stato rimosso l'allora Direttore generale dei Monopoli di Stato, vicenda che aveva interessato anche la Corte dei conti. Questo dirigente, illegittimamente rimosso dall'incarico, naturalmente dovrebbe essere reintegrato ed avere giustizia dopo quanto è intervenuto per legge e per sentenza. È un caso analogo a quello relativo al giudice Carnevale. Riteniamo che il Ministro dell'economia e delle finanze debba dare una risposta su questa vicenda, che richiede appunto soddisfazione. **Sulle

Sin dall'inizio della legislatura, mi sono permesso di chiedere una *par condicio* con la Camera dei deputati in ordine al problema del *question time*.

Quindi, segnalo ai Capigruppo che, qualora volessero chiederlo, si determinerà la diretta televisiva per il *question time*, secondo le modalità previste dal Regolamento. Devo comunque confermare che nessuna richiesta in questo senso è mai stata avanzata dai Capigruppo. Signor Presidente, volevo rilanciare la sua proposta di questa mattina di trovare uno spazio, ma urgentemente, per la conclusione del dibattito sulle questioni comunitarie.